Presidente, poiché non l'ho sentito nella lettura del processo verbale, chiedo che sia inserita nello stesso una frase che si trova a pagina 44 del Resoconto stenografico e precisamente la seguente: «Prima di procedere alla votazione, comunico all'Aula che hanno regolarizzato l'apposizione della firma all'ordine del giorno i senatori Collino, Viespoli, Cursi e Paravia ».

relativamente ad una sua visita di sindacato ispettivo a Rebibbia, dove si è recata a seguito di segnalazioni da parte dell'istituto di reclusione stesso ordine al modo con cui pareva fossero state trattate alcune delle persone arrestate per i fatti di Guidonia della settimana scorsa. A fine seduta affronterò la questione in questi termini. **Discussione

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione esteri ha esaminato in modo approfondito la scorsa settimana il Trattato oggi al nostro esame. La gran parte dei senatori ha convenuto sul carattere storico di questo atto che segna la fine di un lungo contenzioso derivante dal periodo coloniale e pone le basi per un rinnovato sistema di relazioni bilaterali. Solo un Gruppo, l'Italia dei Valori, ha contestato espressamente l'opportunità del Trattato. Questo giudizio negativo è stato anche condiviso dal senatore Perduca, che ha contestato una serie di previsioni in esso contenute, presentando altresì un gran numero di emendamenti che non ha reso possibile la conclusione dell'esame del provvedimento in Commissione. Il principale Gruppo diopposizione, quello del Partito Democratico, attraverso gli interventi della senatrice Marinaro e del senatore Livi Bacci, ha condiviso con i Gruppi di maggioranza la valutazione positiva sul Trattato, che in modo formale sancisce la chiusura di un contenzioso storico; un risultato, questo, cui hanno contribuito diversi Governi negli ultimi 15 anni. In effetti, le premesse del rinnovato stato delle relazioni bilaterali risalgono ai contatti avviati negli anni '90, che hanno condotto al Comunicato congiunto italo-libico del 4 luglio 1998. All'epoca, la Libia era un Paese isolato e l'Italia, con un'azione diplomatica attiva, sentì la responsabilità di ricostruire i rapporti tra la Libia e la comunità internazionale. Grazie in particolare ai nostri sforzi diplomatici, la Libia uscì da quell'isolamento rispondendo alle richieste che provenivano dalle Nazioni Unite, il che portò al superamento delle sanzioni e avviò una normalizzazione dei rapporti diplomatici tra la Libia e i Paesi della comunità internazionale. Con il Comunicato congiunto del 1998, l'Italia espresse per la prima volta il rammarico per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana e, al contempo, espresse l'intenzione di trovare la soluzione di tutti i contenziosi bilaterali e di costruire un rapporto di rispetto reciproco e di collaborazione paritaria. La portata del Comunicato è stata storica e ha messo in rilievo la maturità della democrazia italiana nel riconoscere il proprio passato in una prospettiva realistica. Il Trattato che oggi esaminiamo costituisce il punto di arrivo di lunghe trattative e negoziati che hanno creato le condizioni per il passaggio da quella prima intesa del 1998 ad un vero e proprio Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione. Esso stabilisce che il 30 agosto, anniversario della firma, sia proclamato Giornata dell'amicizia italo-libica. Il Trattato corrisponde agli interessi dell'Italia, ove si consideri la rilevanza della Libia quale *partner* commerciale e interlocutore imprescindibile nel campo della politica energetica, ma anche della disciplina dei flussi migratori in seno al Mediterraneo. Al momento attuale, la Libia rappresenta un'entità a pieno titolo inserita e operante sullo scenario europeo e internazionale e, rispetto all'Italia, vi sono relazioni privilegiate. Del resto, il Mediterraneo e i Paesi della sponda Sud che vi si affacciano sono sempre stati una costante priorità della politica estera dei Governi da oltre vent'anni. Quanto ai contenuti del Trattato, esso si articola in tre Capi. Il primo, dagli articoli 1 a 7, stabilisce i princìpi generali alla base dell'intesa. Si conferma l'impegno delle parti al rispetto della legalità internazionale nel quadro della comune visione di centralità della Carta della Nazioni Unite, cui il Trattato fa continuo riferimento. Vengono poi affermati i princìpi del rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati, del non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza dell'altra parte, della non ingerenza negli affari interni anche impegnandosi, nel rispetto della legalità internazionale, a non usare il proprio territorio in attività ostili verso l'altra parte. Tale impegno, del resto, era già contenuto in maniera succinta nel Comunicato congiunto del 1998. Questa ultima previsione del Trattato è stata oggetto di molti rilievi nel corso del dibattito. In proposito, ribadisco quanto detto in Commissione: non è un patto di non aggressione e non vi è alcuna incompatibilità con il Trattato NATO, qualora la Libia agisca nel quadro della legalità internazionale. È altresì ribadito l'impegno alla soluzione pacifica delle eventuali controversie e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali conformemente agli obiettivi e ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Nel corso dei lavori in Commissione diversi interventi hanno sottolineato la necessità di garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ricordo, signor Presidente, che proprio la settimana scorsa si è svolta in Senato un'iniziativa di celebrazione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ebbene, io credo che, anche in virtù di quanto stabilito dagli articoli 1, 5 e 6 del Trattato, emerga con chiarezza come il rispetto di quanto previsto nei fondamentali documenti su cui si basa la legalità internazionale sia un impegno ribadito nel Trattato che stiamo esaminando. L'Italia dunque potrà sempre richiamare la Libia al rispetto e all'osservanza di questi atti fondamentali senza violare il principio della non ingerenza negli affari interni. Il Capo II (articoli da 8 a 13) reca norme sulla chiusura del capitolo del passato e dei contenziosi ancora in atto. In particolare,l'articolo 8 impegna l'Italia a realizzare in Libia progetti infrastrutturali di base, individuati sulla base di intese bilaterali. Il relativo tetto massimo di spesa complessiva è di 5 miliardi di dollari distribuiti in 20 anni, cioè un importo annuale di 250 milioni di dollari. La Libia renderà disponibili i terreni e agevolerà le imprese esecutrici dei lavori. La realizzazione dei progetti sarà affidata a imprese italiane. I fondi finanziari saranno gestiti dall'Italia e non ci sarà quindi alcun trasferimento di fondi alla Libia. L'articolo 9 istituisce una Commissione mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati, con il compito di individuare le caratteristiche tecniche dei progetti infrastrutturali di base e stabilire la tempistica dei lavori. Tra le iniziative speciali dell'Italia a favore del popolo libico, di cui all'articolo 10, figurano, oltre a quelle già contenute nel Comunicato congiunto(quali l'assegnazione di borse di studio universitarie e post-universitarie a studenti libici,

coloniale), il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici e la costruzione in Libia di 200 unità abitative. Percontro, la Libia, confermando il Comunicato congiunto, si impegna a concedere i visti di ingresso anche ai cittadini italiani espulsi in passato dal proprio territorio che desiderino entrare nel Paese per motivi di turismo, lavoro o altre finalità. Inoltre è previsto, dopo lo scioglimento dell'Azienda libico-italiana, che il fondo speciale da essa costituito sia gestito da un Comitato misto paritetico e destinato alla realizzazione di iniziative speciali, come previsto dal Comunicato congiunto. Ai sensi dell'articolo 13, la Libia e l'Italia si impegnano a raggiungere con uno scambio di lettere una soluzione della questione dei crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti di amministrazioni ed enti libici, sulla base del negoziato finora condotto nell'ambito dell'apposito Comitato misto sui crediti. Nel medesimo scambio di lettere sarà anche definita la questione dei debiti di natura fiscale e/o amministrativa di aziende italiane nei confronti di enti libici. Il Capo III (articoli da 14 a 23) disciplina il nuovo Partenariato bilaterale. Per rinsaldare le relazioni bilaterali già presenti in numerosi settori, le parti costituiscono un Partenariato bilaterale, che si esprimerà attraverso consultazioni politiche su temi bilaterali regionali e internazionali di reciproco interesse. Il Partenariato prevede, tra l'altro, una riunione annuale del Comitato di partenariato, formato dal Presidente del Consiglio dei ministri italiano e dal Segretario del Comitato popolare generale, che si svolgerà alternativamente nei due Paesi. Il Comitato di partenariato adotta i provvedimenti necessari all'attuazione degli impegni previsti dal Trattato. L'articolo 15 prevede un rafforzamento della cooperazione negli ambiti scientifici e della tecnologia, mentre l'articolo 16 è volto ad approfondire la cooperazione culturale e i legami di amicizia tra i due Paesi. L'articolo 17 prevede la collaborazione economica e industriale e l'articolo 18 promuove la cooperazione in materia energetica, di cui le parti si impegnano a favorire il rafforzamento. L'articolo 19 è volto a rafforzare la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina. Per contrastare l'immigrazione clandestina, in base al Protocollo di cooperazione firmato a Tripoli il 27 dicembre 2007, 2007, è previsto il pattugliamento congiunto in mare con equipaggi misti e con motovedette messe a disposizione dall'Italia. È inoltre prevista la creazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane specializzate. Come è stato chiarito nel corso dei lavori in Commissione, si tratterà essenzialmente di un'attività di monitoraggio dei flussi migratori con mezzi satellitari e tecnologici, data la lunghezza e la natura del confine terrestre libico; ciò al fine di individuare provenienza e consistenza delle ondate migratorie e per quanto possibile evitare tragedie umanitarie. Il Trattato prevede altresì una collaborazione nel settore della difesa tra le rispettive Forze armate e tra le industrie militari, oltre a un sostegno alle vittime dello scoppio di mine e alla riabilitazione dei territori libici danneggiati. Con l'articolo 21 le parti si impegnano a collaborare nel settore del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e ad adoperarsi per fare della Regione del Mediterraneo una zona libera da tali armi. Il Partenariato, infine, è esteso allo sviluppo dei rapporti tra i Parlamenti e gli enti locali delle due parti, con l'intendimento di approfondire la conoscenza reciproca. L'articolo 23 reca le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del Trattato e le modalità per le sue eventuali modifiche. Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica, accanto alle consuete disposizioni recanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato, esso reca, all'articolo 3, alcune disposizioni a carattere generale dirette ad introdurre, fino al 2028, un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) residenti in Italia e operanti nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi. Segnalo che da parte della Camera dei deputati è stato aggiunto e approvato un nuovo articolo 4 al disegno di legge di ratifica che reca il riconoscimento di un ulteriore indennizzo a soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Esso dispone, in particolare, l'integrazione delle anticipazioni già percepite da cittadini italiani ovvero da società italiane operanti in Libia a seguito di provvedimenti emanati dalle autorità libiche, ai sensi della legge n. 1066 del 1971. A tal fine il comma 5 dell'articolo 4 istituisce un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dal 2009 al 2011. La Commissione interministeriale per gli indennizzi potrà riesaminare le domande respinte in precedenza per carenza di documentazione. L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento. Signor Presidente,onorevoli colleghi, il Trattato è stato oggetto di un lungo e approfondito confronto sia alla Camera dei deputati sia la settimana scorsa in Commissione. Posso comprendere che siano emersi rilievi su alcuni aspetti di questo Trattato, frutto, come ho detto, di una negoziazione lunga e complessa. Credo tuttavia che oggi il nostro compito sia quello di valutare, al di là delle questioni di dettaglio, il significato politico del Trattato. Su di esso, signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo esprimere un giudizio; un giudizio largamente positivo, ad avviso della maggioranza e di gran parte dei parlamentari dell'opposizione. Siamo il primo Paese ex coloniale che riconosce con chiarezza le responsabilità derivanti dal passato. Questo riconoscimento ci permette di guardare al futuro e di porre così basi solide per un rapporto forte tra le due sponde del Mediterraneo, che deve divenire sempre di più non una barriera, ma un ponte di pace fra culture diverse nella prospettiva di un progresso comune.

è quello molto spesso di tracciare la linea di compromesso tra diritti, o difesa dei diritti, ed interessi, ivi compreso l'interesse nazionale. Appartengo a quella schiera di pensiero politico che non ritiene la parola "interessi" di per sé una mala parola, o una parolaccia, o che pensa, per esempio, che il parlare di interesse nazionale sia di per sé un dato a connotazione negativa; esattamente il contrario.

stiamo parlando di un accordo per sviluppare un rapporto bilaterale speciale e privilegiato attraverso un vero e proprio partenariato, quindi ha un'ambizione che viene ampiamente

democratici pari al nostro. Non è questo il problema, né - ripeto - penso che la difesa degli interessi o dell'interesse nazionale sia di per sé un connotato negativo; al contrario.

che mi sembra configurino non già la soluzione di un lungo conflitto, ma l'apertura di una fase di nuove conflittualità, non solo per la vaghezza di alcune espressioni alquanto rilevanti, per la vaghezza degli strumenti previsti per la soluzione di eventuali conflittualità, nel tralasciare totalmente gli interessi, ad esempio, delle imprese italiane

Credo e temo che, invece di chiudere con il passato, stiamo aprendo una nuova fase di conflittualità, e questo non solo per la personalità della parte contraente.

spesso ambivalente, spesso contraddittoria, ma certamente non confinabile ai dati folcloristici con cui spesso invece si presenta.

infiniti scenari di conflittualità, che sicuramente non possono essere risolti dal puro impegno a dirimerli pacificamente, quando, esattamente in quell'articolo, non si fa riferimento - come spesso si fa né all'arbitrato, né al ricorso alla Corte dell'Aja, ma si rimanda ad una formulazione di «soluzione pacifica». Atti ostili: per esempio, l'attività di opposizione di democratici libici sul territorio italiano è o non è considerabile atto ostile?

che attiene al famoso articolo 13 sui crediti. Le rivendicazioni delle imprese italiane sono quantificate in 620 milioni di euro, ma nulla è detto da questo punto di vista, se non un rinvio ad uno scambio di lettere.

So bene che poi, nel disegno di legge di ratifica, è stato istituito un fondo di 50 milioni di euro, ma non mi pare davvero che questo segni una pagina di svolta, anzi mi pare ne apra di nuove proprio in termini di conflittualità rilevanti.

La controparte è quella che solo la settimana scorsa ha dichiarato e minacciato di non escludere una nazionalizzazione delle proprie riserve energetiche se il petrolio non tornerà a 70 dollari

C'è un rinvio per il 50 per cento a finanziamenti europei non ancora ottenuti, né fissati, né determinati, così come non è quantificato il costo per quanto riguarda le iniziative sociali. Per tutti questi motivi,

fronte ad una controparte che solo una settimana fa incitava tutti i musulmani ad andare a combattere a Gaza; stiamo facendo un accordo con una controparte che solo una settimana fa chiedeva la distruzione dello Stato di Israele; stiamo firmando un accordo privilegiato con una controparte che certamente in termini di evoluzione del rispetto dei diritti non ha un *curriculum* non dico soddisfacente, ma nemmeno di *trend* possibile.

più cogente, più limpido nell'articolato e nella soluzione dei conflitti e più equilibrato rispetto alle parti lese italiane, che pure ci sono.

Tornando indietro di otto mesi, il 29 dicembre 2007 il ministro dell'interno Giuliano Amato e il Ministro degli esteri libico siglarono a Tripoli un Protocollo per la cooperazione tra l'Italia e la Libia per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, mai attuato. Dopo l'accordo firmato dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Gheddafi ha avuto ciò che stava chiedendo dal lontano 1969, anno in cui cacciò solo con le loro valigie i tanti cittadini del nostro Paese che hanno modernizzato il suo Paese. Noi ci troviamo però nell'impellente situazione legata agli sbarchi sull'isola di Lampedusa, dovuti alla negligenza di Tripoli che ha permesso di tutto pur di tenere alta la tensione tra il nostro Paese e la Libia. Ci poniamo delle domande: la Libia vuole davvero bloccare i flussi? La seconda perplessità è se i cittadini del nostro Paese considerino un tale accordo sull'immigrazione sufficiente a giustificare una compensazione nei confronti di un Paese ricco di petrolio. Sono le domande che tanti militanti mi hanno fatto in questi ultimi giorni; domande giuste, lecite, che avranno risposte certe solo quando neanche un barcone approderà sulle nostre coste. Siamo fiduciosi nell'intervento del nostro ministro dell'interno Roberto Maroni, come anche della nostra diplomazia. Il pattugliamento misto dovrebbe portare a risultati concreti, positivi, come già è successo con l'Albania, che con analogo accordo ha totalmente azzerato i flussi migratori verso le coste pugliesi. Ma Gheddafi vuole davvero collaborare con il nostro Paese? Siamo speranzosi, come sempre non ci mettiamo di traverso, siamo fiduciosi nel nostro Ministro. Speriamo solo che tra sei mesi non ci troveremo qui a discutere ancora di sbarchi clandestini dalla Libia: sarebbe un affronto per la nostra gente, uno sgarbo verso il nostro Governo. Sono presenti in tribuna gli studenti dell'istituto "Minucci" di Napoli. Rivolgiamo a loro e ai loro insegnanti, che sono in visita al Senato, il saluto da parte nostra e gli auguri per i loro studi.

colleghe e colleghi del Senato, signori del Governo, la legge di ratifica del Trattato fra Italia e Libia, che questo Senato si accinge a votare, arriva in quest'Aula a meno di un secolo dalla guerra che l'Italia liberale mosse all'Impero ottomano per la conquista di quella che venne battezzata «la quarta sponda». In quella guerra, nella repressione della resistenza autoctona in Cirenaica e in Tripolitania, persero la vita decine di migliaia di persone ed altre decine di migliaia furono vittime di deportazioni ed internamenti. Premetto che molti elementi inducono chi vi parla ad esprimere voto favorevole alla legge di ratifica del Trattato, in conformità col voto espresso dal PD alla Camera e con gli orientamenti del Gruppo in questo Senato. Preminente è il riscatto storico del nostro Paese, che ammette le responsabilità del colonialismo, la cui memoria è rimasta troppo a lungo confinata nelle pagine degli studi degli specialisti. Oggi l'Italia se ne dà ufficialmente carico, e questo è un bene. L'ammissione delle responsabilità comporta anche un risarcimento, il cui prezzo può apparire alto, particolarmente in una fase di grave recessione nella quale finanziamenti vitali sono stati fortemente decurtati. Tuttavia i 5 miliardi di dollari promessi saranno spalmati su venti anni, la gestione dei fondi sarà italiana e le opere iufrastrutturali saranno realizzate da imprese italiane. Ma la normalizzazione dei rapporti con un Paese dalle immense risorse energetiche e con buone potenzialità di crescita potrà alla lunga compensare almeno in parte questi indubbi sacrifici economici. Restano però questioni aperte - sulle quali il Parlamento e la collettività dovranno vigilare attentamente - sui criteri, sulle modalità e sulla correttezza delle procedure nell'espletamento di questo obbligo ventennale. Il Trattato permette di acquisire la Libia allo sforzo della comunità internazionale per il controllo delle migrazioni irregolari. È proprio l'articolo 19 - che sancisce questo impegno cooperativo - che tocca aspetti delicatissimi e controversi ed è su questi che mi voglio brevemente soffermare. Essi configurano le incognite conseguenze di un accordo che contiene rischi che non possono essere sottovalutati e che hanno visto la bilancia del mio personale giudizio incerta nella valutazione di voto, se non mi spingesse al voto positivo la convinzione che le controversie con la Libia vadano chiuse definitivamente. Non sono tanto gli aspetti tecnici dell'accordo a lasciare perplessi, quanto le loro implicazioni. L'articolo 19 conferma i contenuti del Protocollo d'intesa firmato con la Libia a fine 2007, che prevede il pattugliamento congiunto - con unità ad equipaggio misto - delle acque libiche allo scopo di respingere le imbarcazioni con migranti irregolari. L'articolo prevede altresì il finanziamento, con una somma di 150 milioni di euro, di un non meglio definito «sistema di controllo delle frontiere terrestri» libiche, lunghe, come ben si sa, 4.400 chilometri. Si suppone che si tratti di monitoraggio tecnologico (radar, video, sensori e via dicendo) per individuare i flussi in entrata per i mobili e variati itinerari desertici e per permettere una migliore *intelligence* del fenomeno, più che per operazioni di contrasto che non potrebbero essere che sporadiche. In Spagna il sistema SIVE (Sistema integrato di vigilanza esterna), istituito a partire dal 1999, con l'integrazione della sorveglianza elettronica e video con un pattugliamento intensificato, ha permesso di ridurre considerevolmente il traffico di natanti provenienti dal Marocco verso la penisola, prima, e dalle coste africane alle Canarie dopo il 2006. Ma questo effetto positivo non è dovuto solo al SIVE, bensì ad una intensa azione diplomatica volta a concludere accordi di riammissione con il Marocco e con numerosi altri Paesi africani e a sforzi mirati e generosi della cooperazione: un'azione integrata nella quale l'aspetto fisico della difesa dai flussi irregolari è solo parte di un più grande gioco. infatti l'azione meramente fisica di contrasto ha anche effetti negativi: se la sorveglianza si infittisce in una zona, i flussi vengono deviati verso altre, dove i controlli sono minori ma le distanze sono più lunghe, i rischi maggiori; oppure le tecniche di trasporto si adattano, con natanti più piccoli, meno affidabili e più pericolosi, affidandone la guida agli stessi immigrati; o ancora, alzandosi il costo del trasporto o il rischio dello stesso, si selezionano i migranti più disperati o pronti a tutto; oppure, ancora, i tentativi frustrati vengono reiterati. Insomma, ogni barriera può essere aggirata, o valicata, o perforata, al prezzo, magari, di perdite di vite: sono decine di migliaia i migranti morti nei disperati tentativi di navigazione o nelle lunghe marce di avvicinamento ai punti di imbarco. Questo insegna l'esperienza delle migrazioni. Insomma, il contrasto è necessario, ma è solo una componente - e non la più importante - delle politiche migratorie, perché il sistema migratorio è vasto e complesso: i flussi trans-sahariani hanno radici lontanissime nella storia; si valuta che oltre 100.000 migranti si spingano, ogni anno, verso il Nord Africa attraverso molteplici e variabili itinerari; la rete organizzativa di supporto all'immigrazione illegale è ramificata e solida; nei Paesi nordafricani esistono comunità molto numerose di immigrati provenienti dal resto del continente (tra un milione e un milione e mezzo nella sola Libia) che forniscono appoggio e protezione. Inoltre esistono organizzazioni robuste per il traffico degli irregolari capaci di variare ed adattare rapidamente le strategie di trasporto e di inserire nelle loro strategie, mediante la corruzione, coloro che dovrebbero vigilare sui traffici irregolari nei Paesi di origine e in quelli di transito. Le politiche di contrasto, respingimento e rafforzamento dei controlli sono scarsamente efficaci senza robusti accordi di riammissione con i Paesi di origine, che la diplomazia italiana appare meno capace di concludere rispetto a quelle spagnola o francese, e senza robuste politiche di cooperazione, ridotte al lumicino (lo zero virgola zero zero più qualcosa del PIL) nell'anno della Presidenza italiana del G8, ricca di annunci ma povera di risorse. le preoccupazioni maggiori sono di ordine umanitario. L'Europa, e l'Italia con essa, sta tentando una sorta di *outsourcing* delle responsabilità migratorie, spostando sempre più a sud i suoi confini, nel tentativo di proteggere il proprio territorio dagli indesiderati. Se ciò che sta avvenendo a Lampedusa solleva fondatissime critiche (e infatti, come distinguere le posizioni - numerosissime - di coloro che legittimamente chiedono asilo e protezione dalle altre?), le condizioni in Libia sono tremende, come attestato da inequivocabili testimonianze. Per quanto riguarda le condizioni di vita nei campi di detenzione, la sommarietà delle procedure di espulsione, l'inosservanza delle convenzioni internazionali (alcune non sottoscritte), la chiusura del Paese agli osservatori esterni, le denunce delle organizzazioni umanitarie e degli osservatori, della cui imparzialità non è dato dubitare, sono infatti numerosissime e coerenti. Spingere la frontiera a sud significa, per l'Europa e per l'Italia, volgere il capo dall'altra parte sulla sorte di decine di migliaia di migranti, a meno di non pretendere vigorosamente - ma il Trattato è quasi muto in proposito - il rispetto dei princìpi umanitari. Per queste ragioni, un gruppo di senatori del Partito Democratico ha presentato l'ordine del giorno G105, del quale chiedo vigorosamente l'accoglimento da parte del Governo e l'approvazione da parte di tutti i colleghi, col quale si impegna il Governo, in sede di definizione delle intese bilaterali di cui all'articolo 19 del Trattato, ad ottenere garanzie dal Governo libico in tema di rispetto dei diritti umani dei migranti e delle norme del diritto internazionale relativamente alla protezione dei rifugiati. Realismo politico, convenienza e riscatto storico consigliano la firma del Trattato, ma impongono al Governo una *leadership* in Europa per proporre politiche migratorie inclusive, cooperazione rafforzata, rispetto assoluto dei diritti umani. La pagella, per ora, è largamente insufficiente, specie oggi, il giorno successivo alla dichiarazione del Ministro dell'interno (che ci fa rimpiangere un altro Ministro dell'interno del Governo Berlusconi, che aveva ben più coscienza dell'importanza del proprio ruolo)

del Presidente del Senato - una bella e intensa celebrazione del sessantesimo anniversario della solenne Dichiarazione dei diritti umani di fronte a 12 scuole di varie Regioni d'Italia. Grazie!

«ritenendo di chiudere definitivamente il doloroso "capitolo del passato", per il quale l'Italia ha già espresso, nel Comunicato Congiunto del 1998, il proprio rammarico per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana».

quella di tenere viva la memoria del ruolo svolto dai civili e dai militari italiani in quelle zone. Sono stato nominato segretario «per i buoni sentimenti e la giovane età»: così mi è stato detto da persone che hanno mediamente tra gli e che rivendicano la positività della loro esperienza. Ricordo, in particolare, il dottor Leonida Fazi, che venne aiutato nella sua attività di recupero della memoria storica dall'allora direttore de «Il Tempo», dottor Letta.

«Fu giusto o fu sbagliato nulla abbiamo preso, molto abbiamo dato». Questo è lo spirito che voglio qui rivendicare, pur comprendendo pienamente e fino in fondo le ragioni di questo Trattato, ragioni che sostanzialmente condivido

di una verità che va riconosciuta nell'ambito di un Trattato che vuole essere di amicizia per il futuro. L'amicizia si basa infatti sul riconoscimento della verità e sulla condivisione dell'analisi del passato.

il punto di arrivo di un percorso che molto ha impegnato la politica estera italiana e, negli ultimi quindici anni, ben cinque Governi. L'azione dell'Italia e la responsabile mediazione politica e diplomatica svolta hanno convinto Gheddafi ad adempiere alle richieste delle Nazioni Unite, avviando il percorso di normalizzazione dei rapporti tra la Libia ed i Paesi della comunità internazionale e oggi la Libia è un partner economico dell'Italia, in particolare nel settore energetico. II lungo cammino compiuto ha prodotto sicuramente più di un risultato. Il primo è quello di aver fatto uscire la Libia dall'isolamento internazionale e di averla accompagnata in un percorso di normalizzazione nelle relazioni diplomatiche con gli altri Paesi europei e nella costruzione di un vasto sistema di relazioni economiche con l'Europa e gli Stati Uniti, con i quali, in particolare, ha stabilito una forte collaborazione in materia di sicurezza e nella lotta contro il fondamentalismo islamico. Il secondo è quello di aver assolto una nostra responsabilità storica, quella che discende dell'ingloriosa pagina del colonialismo italiano, anche attraverso il lavoro svolto da una commissione mista, da noi sostenuta, per indagare sui conflitti e sui crimini compiuti durante l'occupazione fascista della Libia; siamo il primo Paese ex coloniale che riconosce ed assume la propria responsabilità nei confronti di una ex colonia. Nel lungo negoziato che è stato portato avanti è stata conclusa un'intesa che non è solo italo-libica, ma che coinvolge attivamente l'Unione europea. Infatti, la decisione di costruire un sistema di monitoraggio dei confini libici è parte dell'accordo che la Libia ha stretto con l'Unione europea, prima che con l'Italia, anche in termini di impegno finanziario. Tale valutazione positiva non ci impedisce, però, di vedere i limiti, in particolare in materia di copertura finanziaria e di tutela delle nostre imprese, e i punti critici, che pure ci sono, le problematiche o le difficoltà che devono ancora essere affrontate, tra le quali quella che più di ogni altra inquieta la coscienza di ogni sincero democratico preoccupato della difesa dei fondamentali diritti umani e civili di chi non ha voce né rappresentanza. Perciò anche in quest'Aula, come già alla Camera, con i nostri emendamenti chiediamo che il Parlamento effettui il monitoraggio della complessa esecuzione di tale Trattato e che si intensifichi la pratica degli accordi bilaterali tra l'Unione europea e tutti gli Stati rivieraschi, con un aumento della cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa, che il Governo fa molto male a non finanziare adeguatamente, per dare concreta attuazione ad una politica solidale ed efficace che cerchi di governare il fenomeno degli spostamenti di massa dovuti alla miseria ed alla violenza. Non sono tra quelli che credono che la democrazia sia un bene esportabile, ma tra quelli convinti che solo da una pratica e da una fitta rete di relazioni politiche, economiche, culturali, di scambi e di conoscenza reciproca possa prodursi la contaminazione positiva a cui vanno ascritti i risultati fin qui citati. È un cammino lungo che non si ferma certo alla ratifica di un Trattato ed è un cammino che l'Italia ha fin qui compiuto in virtù del suo ruolo geopolitico di testa di ponte tra Europa ed Africa, ma che non può essere considerato di sua esclusiva responsabilità. D'altro D'altro canto, sarebbe ben strano pensare che un Trattato bilaterale possa risolvere da solo e - come si dice - «qui ed ora» il complesso fenomeno dell'immigrazione clandestina, nonché quello dei flussi migratori che approdano in Italia attraverso le cosiddette aree di transito del Nord Africa. Né si può certo pensare che una problematica di questa portata e di tanta drammaticità possa essere risolta nell'ambito di un rapporto bilaterale e solo nell'area del Mediterraneo, che è un'area di transito, senza prevedere ed attuare una sinergica politica con i Paesi africani. Non si tratta di porre in essere una mera operazione di spostamento dei confini, con il trasferimento delle problematiche note dall'Italia alla Libia, ma di essere in grado di utilizzare ogni piccolo passo in avanti compiuto per costruire le premesse di un'azione multilaterale intesa a definire le forme di collaborazione necessarie a prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori, assicurando gli aiuti allo sviluppo in una prospettiva di pace, sicurezza e valorizzazione della persona. Sappiamo che l'immigrazione proveniente dalla Libia e diretta verso le coste italiane è controllata da organizzazioni criminali, con drammatici costi in termini di vite umane, così come sappiamo che il nostro prossimo obiettivo deve essere quello di annoverare la Libia fra i sottoscrittori della Convenzione di Ginevra sui rifugiati. L'elezione di Gheddafi alla presidenza dell'Unione Africana ci rafforza nella convinzione che la direzione è giusta e che, oggi, possiamo utilizzare tutti gli strumenti politici e diplomatici per ottenere adeguate garanzie da parte della Libia per quanto riguarda i diritti dei migranti e il rispetto delle norme di diritto internazionale, nonché per mettere in atto ogni iniziativa utile affinché le autorità libiche acconsentano allo svolgimento di un'azione di monitoraggio, da parte dell'Alto commissariato per i rifugiati, sulle politiche in materia di immigrazione, con particolare riguardo ai centri di detenzione degli immigrati, aprendo le porte anche alle organizzazioni non governative più rappresentative sul piano internazionale. Tutto ciò considerato, ritengo che opporsi oggi alla ratifica di questo Trattato sarebbe un errore grave e, soprattutto, incomprensibile, non solo per i libici, ma per la comunità internazionale. Valori essenziali come quelli del dialogo, della cooperazione, della sicurezza, della convivenza pacifica hanno bisogno di un largo consenso per poter progredire e produrre risultati misurabili nella vita quotidiana di tutti. Questo è anche il senso degli emendamenti e dell'ordine del giorno che alcuni di noi hanno presentato e che auspichiamo il Governo e la maggioranza abbiano la sensibilità politica di condividere, per dare un senso e una continuità all'impegno comune. A questo fine sollecitiamo il Governo e la Presidenza del Senato a rendere al più presto effettiva la disposizione dell'accordo che estende il partenariato allo sviluppo dei rapporti istituzionali e degli enti locali delle due parti, per allargare la partecipazione e per approfondire la reciproca conoscenza. *(Applausi Grazie!

che chiude - almeno si spera - un vecchio contenzioso con la Libia; un atto che si pone in netta discontinuità con una delle più brutte pagine della storia del nostro Paese e che si spera possa costituire la parola definitiva a non limpide relazioni internazionali tra il nostro Paese e la Libia, che hanno conosciuto nel passato recente anche inquietanti situazioni e risvolti drammatici, e ad atti criminosi non ancora definitivamente accertati. Naturalmente questo lavoro ha potuto prendere corso soltanto quando è cessato il regime sanzionatorio delle Nazioni Unite nei confronti della Libia ed è iniziato - per così dire - un ravvedimento operoso di quel Paese, specie sul fronte della lotta al terrorismo internazionale. Un accordo che guarda, quindi, ad un futuro di relazioni tra i due Paesi, ma anche più in generale tra le due sponde del Mediterraneo, all'insegna di una trasparenza con cui definire una effettiva *governance* per alimentare processi di pace che hanno bisogno di effettivo e convinto sostegno. Un accordo che potrebbe costituire un modello di relazioni con cui avvicinare le due sponde, che conoscono da decenni dinamiche divergenti e confliggenti. Ne sono dimostrazione le opposte dinamiche demografiche, così come quelle economiche e sociali. Processi che hanno conosciuto negli anni recenti flussi migratori non controllati e che il Trattato in questione vorrebbe avviare a soluzione. È risaputo infatti che il Governo libico, periodicamente, quando vuole mettere sotto pressione il Governo italiano, dà il via libera agli sbarchi di clandestini. Numerosi sono gli emigranti che stazionano sulle coste libiche in attesa di un imbarco di fortuna. Ma questo è un accordo rilevante anche dal punto di vista del partenariato energetico e industriale; dunque, per un Paese come il nostro, che ha bisogno di diversificare le proprie fonti energetiche, è certamente molto importante. Come, del resto, gli elementi che guardano agli interventi significativi di realizzazione infrastrutturale costituiscono un aspetto di sicura importanza per un Paese come la Libia non solo dal punto di vista del risarcimento storico. Con tutto ciò non possono essere sottaciuti elementi di pesante ambiguità che permangono nell'accordo e che gettano perplessità sull'intera operazione politica e diplomatica. Aspetti che evidentemente richiedono, da un lato, un attento monitoraggio circa il rispetto delle clausole contenute e, dall'altro, una maggiore chiarezza interpretativa, come nel caso delle clausole in cui siprevede una sorta di indisponibilità del nostro Paese ad utilizzare il proprio territorio per iniziative contro la Libia; clausola che evidentemente mal si concilia nel caso in cui l'azione fosse mossa o richiesta da organismi internazionali di cui facciamo parte, come la NATO, e che vincolano il nostro Paese al rispetto di quei patti senza limitazione o eccezione territoriale alcuna. Il Trattato prevede anche il controllo e un pattugliamento delle coste da parte della Marina italiana assieme alla Marina libica ed un controllo delle frontiere terrestri della Libia. Anche su questo punto il Trattato contiene elementi di ambiguità. Il problema dei confini meridionali della Libia non è semplice. C'è il rischio - come è stato ricordato da molteplici interventi, anche nel dibattito alla Camera - che il controllo delle frontiere libiche si possa effettuare con il nostro coinvolgimento in azioni sulla frontiera che ci potrebbero mettere in grande difficoltà, stante la situazione di forte criticità cui la Libia è sottoposta dagli organismi internazionali, specie per quanto riguarda appunto le frontiere meridionali. L'Italia, oltre a presentare le sue scuse e a rendere omaggio alla memoria e alla storia libica, garantisce il versamento di 5 miliardi di dollari in venti grosso modo la stessa entità delle misure anticrisi con cui si rifinanzia la legge obiettivo (questo detto per inciso). Si impegna poi per la realizzazione di un'autostrada costiera di oltre 1.600 chilometri, che unirà la Libia alla Tunisia da una da una parte e all'Egitto dall'altra, per la costruzione di 200 abitazioni, per un progetto di sminamento del Paese, per il finanziamento di borse di studio a studenti libici e per le pensioni ai mutilati dalle mine piazzate dagli italiani in epoca coloniale e agli ascari che combatterono durante la Seconda guerra mondiale nelle file dell'esercitoitaliano. Tutto ciò costituisce un gravoso impegno finanziario assunto dall'Italia in un momento in cui, tra l'altro, il Governo ha operato tagli rigorosi al settore della cooperazione internazionale. Al riguardo, il Governo è sicuro di aver fornito la necessaria e prevista copertura finanziaria al provvedimento o invece, come è stato detto e scritto, si ricorrerà ad un'addizionale energetica da parte dell'ENI? UnTrattato poco trasparente che si propone trasparenza non è di per sé molto convincente. Eppure, nonostante questo, è necessario investire nella fiducia e nel futuro tra tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ma se non si vuole che la fiducia per un futuro di pace e di benessere possa rappresentare solo un'effimera speranza occorre investire operativamente affinché quei presupposti si realizzino davvero e, per farlo, occorre che l'attività di vigilanza del Parlamento costituisca il fulcro di un monitoraggio continuo al Trattato e alla sua rigorosa interpretazione e applicazione. Questo credo sia legittimo chiedere e pretendere, affinché gli elementi di ambiguità ancora persistenti si diradino e il Trattato siglato con la Libia possa davvero costituire per il futuro un esempio fulgido per affrontare e risolvere i problemi legati al governo dei flussi migratori e allo stesso tempo costituire occasione di sviluppo. Solo in questo senso sarà da auspicare l'estensione di un suo modello applicativo per affermare un modello di relazioni internazionali multilaterali non più solo nell'ottica di rapporti e accordi bilaterali.

di legge n. 1333** Cari colleghi, più volte nell'ambito della discussione generale che si sta svolgendo da questa mattina ho sentito definire il Trattato di amicizia con la Libia come un atto fondamentale che ricuce gli strappi nella storia, che risana le ferite operate dalla politica estera italiana negli anni più neri del nostro percorso nazionale. Tante volte ho sentito dire che l'eredità colonialista, il fardello che pesava sul nostro futuro di Nazione democratica e pacifica, sarebbe stato tolto con la conclusione dell'Accordo al quale hanno lavorato da anni i nostri Governi. Troppe volte, potrei dire, ho sentito cantare, come ne «La Ginestra» di Leopardi, le «magnifiche sorti e progressive» che il Trattato avrebbe permesso di conseguire, troppe per non pensare alle parole con le quali il Leopardi

la confusione che contraddistingue la discussione sviluppatasi attorno al Trattato parte da un assunto fondamentale, che sembra abbiate dimenticato: se l'eredità colonialista vuol esser cancellata, allora è con gli aiuti a quel popolo che tempo addietro soggiogammo che dovremmo farlo, non con un Trattato che premia *in primis* il governo libico e, subito dopo, le imprese italiane che riceveranno benefici economici dalla sua entrata in vigore! Si sarebbe dovuto chiudere il capitolo con un Trattato aperto e dibattuto dal Parlamento, luogo sovrano delle decisioni. Si sarebbe dovuto scrivere il capitolo finale con un Trattato che, nel sanare i conflitti nati dal colonialismo, dispone anche affinché mai più nessun tipo di colonialismo possa svilupparsi, neppure nella forma «dolce» del neocolonialismo economico, ossia quella forma di imperio economico che spinge i migranti dai Paesi più poveri a rischiare la vita questo Trattato ricomprende i vizi ma non le virtù. Iniziando dal percorso che ha portato alla ratifica di oggi. Un percorso che alcuni potrebbero definire come caratterizzato da discrezione diplomatica. Ma la discrezione, vi ricordo, quando riguarda la cosa pubblica, diventa omissione di informazione alla pubblica opinione. Perché il testo dell'Accordo è diventato di pubblico dominio con cinque mesi di ritardo dalla firma apposta a Bengasi, il 30 agosto 2008, e cioè soltanto quando è stato calendarizzato in discussione alla Commissione affari della Camera in data 13 gennaio 2009. Nel vuoto intercorso abbiamo appreso le notizie circa la dimensione dell'impegno economico, la differente formulazione del testo nella versione libica ed in quella italiana, e la problematica della cosiddetta ENI-*tax* soltanto da fonti giornalistiche. E anche stamani, cari colleghi, questa discussione generale è una discussione monca, dato che ci possiamo esprimere soltanto sul disegno di legge di ratifica, che consta di soli sei articoli, caratterizzati da formalismo in quanto attinenti per lo più alla copertura economica degli impegni bilaterali presi, e nulla possiamo aggiungere al contenuto del Trattato stesso, il cui articolato, ben più ampio e pregnante, si riferisce invece alla sostanza degli impegni presi. La stessa considerazione è stata da me mossa in Commissione affari esteri, ed anche il sottosegretario Mantica ha convenuto che, inizialmente, il proposito del Governo era quello di scindere la ratifica parlamentare dalla introduzione delle disposizioni contenute nel disegno di legge medesimo in due provvedimenti distinti. Non voglio Non voglio con questo scardinare la prassi invalsa per la quale i Trattati internazionali sono materia del Governo e non dell'opposizione, ma voglio dire che se si fosse mantenuto un livello più alto di coinvolgimento della stessa opposizione della pubblica opinione, e non si fosse chiuso ad agosto, in fretta ed in segretezza, un percorso sviluppatosi per anni con continue mediazioni, forse non ci ritroveremmo oggi, come Italia dei Valori,

Permettetemi dunque, dopo aver dato conto della forma, di entrare nella sostanza dell'Accordo. Innanzitutto vorrei esprimere il disagio che provo nel constatare come nel testo dell'Accordo manchi *in toto* la predisposizione di meccanismi di tutela dei diritti umani. Non basta, come mi è stato risposto in Commissione, il generico riferimento fatto dal Trattato all'articolo 6 circa il rispetto dei princìpi delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale universale dei diritti dell'uomo, in quanto se i diritti dichiarati non vengono sostanziati ed implementati da provvedimenti specifici, rimangono solo vuoti intenti. Da fonti ufficiali, risulta indubbio che la garanzia dei diritti universali dell'uomo non raggiunge gli *standards* di un Paese democratico, e tante sono le storie degli immigrati subsahariani respinti alle frontiere, ricacciati nel deserto, abbandonati. Tramite il Trattato in discussione l'Italia avrebbe potuto impegnare la Libia a fornire meccanismi di tutela ed assistenza ai migranti; avrebbe potuto invitare Gheddafi a ratificare la Convenzione Onu sui diritti umani avrebbe potuto istituire un sistema di costante monitoraggio, anche tramite ONG specializzate, sul trattamento riservato a tali immigrati; avrebbe potuto, infine, spingere affinché nell'ordinamento interno libico venisse introdotto lo strumento dell'asilo politico per coloro che provengono da territori segnati da guerre e regimi dittatoriali. Ma lo spirito con cui il nostro Governo si è mosso non è stato quello di creare una zona di democrazia e di Stato di diritto, quanto quello di erigere un muro che bloccasse gli immigrati prima della frontiera italiana, perché, si sa, quello che poi ha un ritorno elettorale in sostanza è la lotta «dura» e miope, ossia sul breve periodo, ai clandestini! E allora ai clandestini! E allora ritorno alle premesse iniziali, cari colleghi, quando dicevo che per chiudere il capitolo del colonialismo si dovrebbe porre le basi per scongiurare qualsiasi forma di colonialismo per il futuro, A fronte di un impegno dell'Italia e dell'Unione europea, non si riscontra alcuna contropartita per il governo libico in termini di clausole per la salvaguardia dei diritti dei migranti. Consideriamo, dunque, il tema dell'impegno economico che tale Accordo pone all'Italia, e valutiamone il valore in ottica comparata rispetto alle manovre approntate per far fronte alla crisi: il Trattato di amicizia prevede per Gheddafi la somma di 5 miliardi di dollari, mentre per sostenere i cittadini italiani ne impegniamo, con il cosiddetto decreto anticrisi, soltanto 4 di miliardi. Non si può non scorgere nell'impianto generale una certa miopia.

Per ciò che attiene all'inserimento del Trattato nel sistema giuridico internazionale, sussiste un *fumus* d'incompatibilità fra gli impegni presi ad agosto tramite il Trattato di amicizia con la Libia e quelli sanciti nel 1949 con la ratifica del Patto atlantico. In particolare, l'Italia si astiene da qualsiasi forma di ingerenza diretta o indiretta negli affari interni ed esterni dell'altro Paese e dichiara che non userà, né permetterà, l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro la Libia. Invece, l'articolo 5 del Patto atlantico enuncia che le parti concordano che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o in America settentrionale, deve essere considerato come un attacco contro tutte e di conseguenza concordano che, se tale attacco armato avviene, ognuna di esse, in esercizio del diritto di autodifesa individuale o collettiva, riconosciuto dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti attaccate prendendo immediatamente, individualmente o in concerto con le altre parti,

detto articolo, che l'Italia metta a disposizione della Libia le nostre tecnologie *radar* per vigilare sulle frontiere di terra del Paese, ossia quelle interne. Tale disposizione potrebbe essere anche meritoria, in quanto permette di controllare i flussi in arrivo di migranti e di gestirli in maniera positiva. Tuttavia ritorna, subito, la considerazione fatta sull'assenza di garanzie del rispetto dei diritti fondamentali.

l'Italia prevede di partecipare soltanto al 50 per cento, cioè con 152 milioni, demandando il resto dei finanziamenti all'Unione europea sulla base - si legge nel testo Intese a suo tempo intervenute tra la Grande Giamahiria e la Commissione Europea». Avevo chiesto in Commissione se il Governo ritenesse corretto impegnare l'Italia in un progetto senza sapere se realmente l'Europa sarà davvero un co-finanziatore, col rischio di una mancanza di copertura finanziaria e di una ingerenza nelle politiche europee delle quali ovviamente non possiamo dettare autonomamente l'agenda. Il sottosegretario Mantica mi ha risposto che gli accordi europei sono in via di definizione nelle competenti sedi europee. Ma allora torno a domandare al Governo: al Governo: le intese sono intervenute a suo tempo, come si legge nel Trattato, o sono in via di definizione, come afferma il Sottosegretario? Il Parlamento necessita di una risposta seria e precisa!

Ebbene cari colleghi, ho il fondato timore che proprio questo il Governo abbia fatto firmando il Trattato, e proprio questo, ossia retrocedere fingendo di andare avanti, il Parlamento si appresti a fare se

È veramente molto spiacevole. Tuttavia, voglio dare l'ennesima fiducia a questi Governi libici, che non hanno fatto niente finora per risolvere i problemi dei cittadini libici, di questi poveri disgraziati che continuano ad arrivare da noi in cerca di una vita migliore. Nell'annunciare l'apertura del CIE a Lampedusa, il ministro Maroni ha dichiarato che il Ministero sta avviando le procedure affinché in poco tempo si completino i primi rimpatri da Lampedusa di tutti gli immigrati, ad esclusione dei minori. Infatti, oggi da Lampedusa partiranno i primi immigrati per ritornare a casa, finalmente. *(Applausi dal Gruppo LNP).* Invece di pensare a presentare emendamenti per questi poveri disgraziati, iniziate a presentare emendamenti anche per i poveri vostri paesani, per il vostro popolo! No. Bugiardo sarai tu, non io! Le polemiche sull'apertura di questo nuovo centro di identificazione e di espulsione sull'isola

Io ho l'isola sottosopra per colpa vostra, perché non avete saputo dare le informazioni giuste. Il progetto del Governo e del ministro Maroni è ottimo. Andrà avanti. L'ho sposato subito perché questo fenomeno lo voglio eliminare. Questi poveri disgraziati che continuano a sbarcare nella nostra terra in cerca di una vita migliore non fanno altro che andare nelle strade perché noi come voi in passato non abbiamo saputo gestire questo fenomeno. Noi finalmente oggi riusciremo a farlo perché i trafficanti di uomini devono sapere che arriveranno a Lampedusa e ritorneranno a casa. Chi può andare a casa deve farlo: questo è ciò che ci importa, perché personalmente voglio pensare soprattutto ai problemi che affliggono da vent'anni ormai la mia isola e che sono problemi seri. Voi lo sapete: nell'isola di Lampedusa mancano tanti servizi. Come facciamo a dare ospitalità a questi poveri disgraziati se neanche li possiamo ospitare? Quindi, il progetto del ministro Maroni è ottimo. Ci vorrebbero altri uomini così decisi e fermi come il ministro Maroni proprio per salvare soprattutto questi poveri disgraziati che si imbarcano in quelle carrette e arrivano da noi e arrivano da noi senza nessuna speranza. Questa è l'unica cosa vera, cari colleghi, di sinistra soprattutto, perché siete voi che in questi mesi e in questi anni avete dato loro la possibilità di venire nella nostra terra e di...

ed è vergognoso che ancora, dopo tanti anni, il nostro Governo debba pagare. Quindi, il nostro popolo ha scelto noi e deve confidare in noi perché noi libereremo il nostro Paese da questo brutto fenomeno!

*(PD)*. Signora Presidente, cari colleghi, altri senatori del mio Gruppo hanno già motivato le ragioni del nostro voto favorevole

che in questa discussione verifichiamo una questione che riguarda in generale la linea di condotta - vero, presidente Dini? - della nostra politica estera, cioè la capacità

affermato: interesse nazionale e princìpi non possono essere contrapposti. Naturalmente, dobbiamo sapere che non si tratta di una disquisizione teoretica. Questo tentativo di trovare un equilibrio tra il realismo politico e i princìpi, tra quelle ragioni che ci spingono all'approvazione dell'Accordo e i motivi di preoccupazione, che peraltro sono emersi in modo ampio nella nostra discussione, si svolge si svolge in uno scenario drammatico che ha le caratteristiche di una vera e propria tragedia biblica e cha riguarda migliaia di persone ed ha portato molte di loro a perdere la vita. Si tratta pertanto di una questione di enormi dimensioni e io non sarei a posto con la mia coscienza se non dicessi che tali preoccupazioni non riguardano solo l'atteggiamento, la storia e le posizioni del Governo libico, ma anche le nostre difficoltà di di trovare un punto di equilibrio convincente fra il contrasto all'irregolarità dell'immigrazione e il rispetto intransigente dei diritti umani ed una capacità di apertura alle persone. È per questo, credo, sottosegretario Mantica, non solo per una riserva, riserva, che pure può esistere nei confronti di molti atteggiamenti del Governo libico, ma per un bisogno di verificare noi, passo per passo, la nostra capacità, quella del Governo italiano e delle forze politiche di essere all'altezza, nei loro comportamenti pratici delle affermazioni che pure compiono dal punto di vista politico generale, è per questo, dicevo, che abbiamo bisogno di una forte azione di monitoraggio e di verifica, di

le conseguenze degli atti che compiamo e ad assumerci nel tempo la responsabilità di una verifica e, naturalmente, anche di una messa a punto, nelle nostre scelte, delle azioni conseguenti. Questo è quanto volevo dire. Per tale ragione abbiamo presentato,

*(PdL)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, illustre sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Mantica, i trattati internazionali rappresentano sempre un'importante pagina di storia, in particolare quando, come nel caso in esame, chiudono una dolorosa pagina del passato per aprirsi alla speranza del futuro. Il Trattato sottoscritto il 30 agosto 2008 dal presidente Berlusconi con la Libia chiude un periodo di risentimenti e di rivendicazioni e ne apre uno nuovo, di collaborazione e pacificazione. Dal prossimo anno, infatti, in entrambi i Paesi sì celebrerà, il 30 agosto, la «Giornata dell'amicizia» e cesserà conseguentemente in Libia la «Giornata della vendetta». Tra le disposizioni del Trattato assumono particolare importanza quelle recanti l'impegno della Libia a concedere i visti di ingresso per motivi di turismo, lavoro o altre finalità anche ai cittadini italiani espulsi in passato dal territorio libico, nonché quelle concernenti l'impegno a definire le pendenze in ordine a crediti e debiti fiscali e/o amministrativi di aziende italiane. L'Accordo è finalizzato quindi ad instaurare un rapporto diverso nelle relazioni tra Italia e Libia e ad intensificare la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina ed irregolare, mediante un pattugliamento delle coste da parte della Marina italiana insieme alla Marina libica, intervento quest'ultimo quanto mai attuale e necessario al luce del persistere di flussi migratori clandestini di provenienza libica. Sarà anche migliorata la collaborazione nel settore difesa nell'ottica della non proliferazione degli armamenti e del disarmo. Il disegno di legge individua le misure finalizzate alla copertura finanziaria degli interventi previsti nel Trattato, in particolare quelli di carattere infrastrutturale, mediante una addizionale IRES a carico dei soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, per venti anni, cioè fino al 2028. Altre disposizioni, parimenti importanti, sono volte al riconoscimento di un ulteriore indennizzo che chiude definitivamente la fase risarcitoria ai soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Il Trattato fissa al Capo I i princìpi generali dell'accordo e precisamente: l'impegno reciproco al rispetto della legalità internazionale; l'uguaglianza sovrana; il non ricorso alla minaccia e all'uso della forza; la non ingerenza negli affari interni; la soluzione pacifica delle controversie; il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; la promozione di iniziative volte a favorire il dialogo e la comprensione fra i due popoli. Il Capo II reca disposizioni volte a sanare le situazioni pregresse e i contenziosi pendenti fra i due Paesi. Di particolare interesse sono le norme contenute nell'articolo 8 che impegnano il nostro Paese a realizzare in Libia un programma infrastrutturale ventennale: una grande occasione, un nuovo mercato per le nostre imprese. Un vero e proprio mercato parallelo in un momento di gravissima crisi in cui il rilancio delle infrastrutture rappresenta una priorità del Governo per la ripresa dell'economia. Tali infrastrutture saranno individuate da una commissione mista paritetica, su proposta della Grande Giamahiria, con una copertura finanziaria garantita da fondi reperiti e gestiti dal nostro Paese per un importo complessivo di 5 miliardi di dollari USA, con un impegno annuale quindi di 180 milioni di euro, e saranno realizzate esclusivamente "esclusivamente" - da aziende italiane su siti resi disponibili dalla Libia, senza oneri per l'Italia e le stesse ditte esecutrici, in conformità a specifici cronoprogrammi. L'Accordo prevede altresì agevolazioni in favore delle aziende per favorire il reperimento dei materiali da costruzione, l'espletamento delle procedure doganali e di importazione e la fruizione di taluni servizi (energetici e telefonici). La Libia si impegna inoltre a garantire, a seguito di trattative dirette con aziende italiane, la realizzazione di opere, progetti industriali ed investimenti nel proprio territorio, nell'ottica di una forte cooperazione

L'articolo 10 pone a carico del nostro Paese talune iniziative speciali in favore del popolo libico, sulla base di specifiche richieste libiche, da finanziare con il Fondo sociale istituito ai sensi dell'articolo 12 del Trattato. Si tratta di borse di studio universitarie e postuniversitarie; di programmi di cure presso istituti specializzati italiani in favore di vittime dello scoppio delle mine; del ripristino del pagamento delle pensioni di guerra; della restituzione di reperti archeologici e di manoscritti. Si segnala, tra le predette iniziative speciali, la costruzione di 200 unità abitative in Libia, su siti e con caratteristiche da determinare di comune accordo. Il Capo III reca la disciplina del nuovo partenariato bilaterale con previsione di consultazioni politiche a vari livelli su temi bilaterali, regionali e internazionali, di reciproco interesse. Il Comitato di partenariato, inoltre, adotta i provvedimenti necessari all'attuazione degli impegni previsti dal Trattato. Altre disposizioni del Capo III attengono al rafforzamento della cooperazione fra i due Paesi in diversi campi di comune interesse, come quello scientifico, tecnologico, medico-sanitario e culturale. Norme specifiche sono poi volte a favorire la collaborazione economica, industriale ed energetica, anche attraverso la promozione di progetti di trasferimento di tecnologie. Riveste particolarmente importanza la collaborazione nei settori delle opere infrastrutturali dell'aviazione civile e delle costruzioni navali, anche attraverso la costituzione di società miste, la promozione di iniziative di sostegno delle piccole e medie imprese e l'incentivazione degli investimenti diretti. Alla luce di quanto esposto, ritengo sia evidente che, accanto ad una giusta ed equa finalità risarcitoria e all'apertura di una nuova fase storica di collaborazione e cooperazione fra i due Paesi, emerga un altrettanto importante e strategico risultato del Governo: un nuovo mercato in Libia, esclusivo per le nostre imprese, per un periodo di ben venti anni, con un investimento complessivo di ben 5 miliardi di dollari USA. Siamo di fronte, quindi, a decisi interventi che incideranno favorevolmente sull'economia italiana con investimenti infrastrutturali importanti che non ricadono come si è già avuto modo di illustrare - direttamente sul bilancio dello Stato e che si affiancano a quelli previsti nel decreto anticrisi, da poco approvato in Senato. Ritengo che i risultati raggiunti dal presidente Berlusconi con il Trattato in discussione siano da ritenere di portata storica, così come peraltro ribadito dal presidente Dini nel suo intervento introduttivo, e debbano perciò essere tenuti in grande considerazione, ancor più in questo momento di grande difficoltà internazionale. Concludo dichiarando il mio voto favorevole. Signora Presidente, mi sono un po' vergognato, come si vergognò Montanelli quando dinanzi ad alcune affermazioni, lesive del nostro Paese, disse che è un fenomeno ricorrente in Italia parlarci male addosso e definì questi fenomeni espressi da italioti.

occupante inglese, dopo la sconfitta del 1945, riconobbe durante il suo mandato che l'Italia aveva fatto opera di civiltà in Libia e quindi auspicava - il nemico inglese - che ci fosse dato anche il mandato, come l'avemmo poi per la Somalia. Qui invece si parla di vergogna, di di inenarrabili delitti da noi commessi; però, nello stesso tempo, nel Trattato si dice che riconosciamo la pensione ai combattenti libici, quelli che combatterono fino all'ultimo momento con noi. Allora, credo che qualche italiota qua dentro dovrebbe visitare la Libia per vedere quello che il Governo italiano aveva fatto. Altro che delitti commessi! Opera di civiltà. Adesso porteremo pure il caffè al beduino sotto la tenda; ma quelli restano sempre coloro che evirarono i nostri prigionieri a Shara Shat e a cui tagliuzzarono le labbra e la lingua perché non potessero bere, perché morissero di sete. Questa è la civiltà di quel popolo che noi avremmo martoriato. Questi non hanno mai capito nulla della grande civiltà di Roma che noi fummo capaci di portare in terra di Libia. Quindi, italioti che oggi avete preso la parola, siete italioti.

*(PD)*. Signora Presidente, come ho detto stamani, vorrei denunciare la campagna che è stata lanciata contro l'onorevole Bernardini e l'ex onorevole D'Elia, a seguito della loro visita ispettiva al carcere di Rebibbia, dove si erano recati a seguito di segnalazioni per cercare di capire cosa fosse in effetti successo a due dei romeni accusati dello stupro di Guidonia della settimana scorsa. Senato su quanto avvenuto di lì a poco, cioè sabato scorso durante la trasmissione «Effetto sabato». Ebbene, un certo signor Maurizio Battista, che mi si dice essere un comico, senza alcun tipo di contraddittorio e con l'appoggio esplicito della stessa conduttrice, ha sottoposto a pubblico dileggio la visita dell'onorevole Bernardini e dell'ex onorevole D'Elia e ha travisato completamente il motivo di quella visita. Infatti appunto, come è stato detto, i due si erano recati in carcere per cercare di capire ciò che era successo. Le frasi del signor Battista sono drammatiche e avvengono in un contesto che dimostra, ancora una volta, che il nostro servizio radiotelevisivo non è sotto controllo. Mi domando, se il Senato ritiene di doversi unire nell'espressione della solidarietà all'onorevole Bernardini e all'ex onorevole D'Elia che hanno ormai la casella di posta elettronica intasata di messaggi minatori, in particolare rivolti all'onorevole Bernardini con argomentazioni non dissimili da chi ha praticato lo stupro nei confronti delle vittime di Guidonia, e se non sia anche il caso di avviare un dibattito relativamente al modo con cui i nostri mezzi di comunicazione stanno coprendo qualsiasi cosa avvenga o non avvenga

a quella vicenda possa contribuire a far sì che nelle prossime settimane episodi di questo tipo, vista e considerata la grancassa mediatica, divengano una triste quotidianità per questo nostro Paese. Signora Presidente, intervengo in merito a questo ultimo intervento dell'onorevole Perduca per sottolineare un fatto veramente grave rappresentato dalle accuse che alcuni parlamentari hanno rivolto agli operatori delle Forze di polizia che hanno arrestato gli autori di gravissimi reati. Vede, l'onorevole Sergio D'Elia, condannato per l'omicidio di un poliziotto senza aver mai risarcito risarcito il danno alle vittime, non si può presentare in un istituto di pena per fare delle accuse nei riguardi delle forze dell'ordine e delle istituzioni di questo Paese. Caro senatore Perduca, sbagliate quando fate questo tipo di attacchi nei riguardi delle istituzioni del nostro Paese... PERDUCA. Quali No, senatore Perduca, lei ha potuto svolgere il suo intervento senza interruzioni. Lasci svolgere l'intervento al senatore Saltamartini! SALTAMARTINI *(PdL)*. Non potete dare lezioni...

Dopo di che, c'è un giudice nel nostro Paese che potrà giudicare quello che voi sostenete. Ma sono trent'anni che le Forze di polizia stanno ad ascoltare le vostre aggressioni. Lei la deve smettere, senatore Perduca! E, soprattutto, chi si è reso responsabile - lo ripeto - di aver ammazzato un ragazzo di vent'anni senza aver mai chiesto scusa alla sua famiglia, né aver mai risarcito il danno, non può dare lezioni di moralità, né in quest'Aula parlamentare, né nel nostro Paese. Presidente, con pacatezza: nessuno ha accusato gli agenti di polizia di aver fatto un pestaggio. Anzi, proprio per verificare

quelli che difendono gli stupratori e che accusano ingiustamente gli agenti di polizia penitenziaria. Non esiste uno schieramento del genere.

a trovare e portare solidarietà alla famiglia e a quella coppia che ha subìto una violenza e che resterà a vita marchiata, e non persone che hanno violentato e che avevano già premeditato violenze in precedenza. Chi andate a visitare? I carnefici. *(Commenti dei senatori

a trovare le persone che hanno subìto una violenza. È inaudito pensare che l'onorevole Bernardini si lamenti delle minacce ricevute per essere andata a trovare una persona che ha violentato

apre una nuova finestra"). Colleghi, comunico che, d'intesa con il Presente della Camera dei deputati, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è convocata per domani, mercoledì 4 febbraio 2009, alle ore 14, presso la sede di Palazzo San Macuto per procedere alla propria costituzione. **Interpellanze